il provvedimento che ci ritorna dalla Camera contiene modificazioni di tutto rilievo anche e soprattutto in materia fiscale. Segnalo innanzitutto che all'articolo 15 si è disposto il mandato al Governo per l'approvazione, entro il 31 dicembre 2013, di norme che rendano stabili gli incentivi fiscali e cioè che essi si applichino, con aliquote da determinare, per un periodo ben superiore Inoltre è stato aggiunta, sempre dalla Camera, l'ulteriore fattispecie concernente l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico a cui, quindi, competono, nei limiti consentiti, sia le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, sia quelle previste dall'articolo 16 per interventi di ristrutturazione edilizia. Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 15 prevede che con ulteriori provvedimenti, da emanare entro il 31 dicembre 2013, va presa in considerazione l'opportunità di agevolare ulteriori interventi nel settore dell'edilizia quali, ad esempio, le schermature solari, la sostituzione dell'amianto con materiale non inquinante ed altri interventi minori. All'articolo 16 è stato aggiunto il comma 1-*bis*, con cui viene concessa la detrazione del 65 per cento anche per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici ubicati in zone ad alta pericolosità sismica indicate da provvedimenti già in essere. È stato introdotto un nuovo articolo, il 16-*bis*, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze promuova, di concerto con l'ABI, una verifica delle condizioni che gli istituti di credito offrono ai soggetti che intendono avvalersi dei benefici fiscali, sia per interventi di efficienza energetica, che per quelli di ristrutturazione edilizia, per finanziare le opere necessarie per tali interventi e servizi. All'articolo 19 vengono introdotte significative modificazioni relative all'aumento dell'IVA, dal 4 al 21 per cento, per i prodotti editoriali a cui sono allegati supporti integrativi. In particolare, viene chiaramente definito cosa si deve intendere per supporto integrativo, e cioè i nastri, i dischi, le videocassette, altri supporti sonori, videomagnetici o digitali, che l'aumento anzidetto dal 4 al 21 per cento non si applica ai supporti ceduti, anche gratuitamente ed in un'unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado, per le università e per i libri fruibili dai disabili visivi. Ulteriore condizione è che i prodotti editoriali di cui innanzi abbiano un prezzo indistinto e non siano commercializzabili distintamente. Rammento che le indicate norme hanno effetto dal 1° gennaio 2014. Con queste nuove norme si è data piena attuazione all'ordine del giorno approvato a maggioranza totalitaria da questo Senato con cui si chiedeva la non applicazione dell'aumento dell'IVA, guarda caso, ai supporti integrativi di prodotti editoriali per le scuole e i disabili. L'articolo 21, relativo alle disposizioni

sono state introdotte ulteriori modifiche, in particolare alla prima parte del provvedimento, dall'articolo 2 all'articolo 7, che è concentrata nel recepire la direttiva comunitaria n. 31 riguardante la prestazione energetica nel settore dell'edilizia. In particolare, sono state modificate alcune definizioni allargandone il senso e il significato, soprattutto in riferimento ai concetti di energia esportata, di fabbisogno annuale globale di energia primaria, di impianto termico allargato alla definizione di impianti tecnologici. Si fa inoltre riferimento alla necessità che il Ministero dello sviluppo economico si possa avvalere della competenza dell'ENEA nell'emanazione dei decreti relativi alle modalità di progettazione per i suddetti impianti.

per i cosiddetti edifici ad energia quasi zero, introducendo la necessità di tenere in debita considerazione l'esigenza prioritaria, da tutti condivisa, del contenimento del consumo di territorio.

le nostre obiezioni e le nostre valutazioni critiche. Mi riferisco in particolare all'introduzione di una clausola di nullità dei contratti di vendita nonché dei contratti riferiti al trasferimento di immobili a titolo gratuito e degli stessi nuovi contratti di locazione ove non vi fosse allegato l'attestato di prestazione energetica.

dell'impatto del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali: una sorta di monitoraggio che credo possa essere utile, e che condividiamo,

Questo atto del Senato è la prova provata che noi siamo in grado di apportare idee e contributi nell'interesse generale del Paese e rispetto ai problemi reali che lo attraversano.

a prevedere iniziative dirette a dare stabilità alle agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici, attualmente previste in misura pari al 65 solo fino al 31 dicembre 2013, così da permettere il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020, e a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui in tema attraverso interventi diretti a favorire l'accesso al credito per misure di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia. Siamo noi che qui riproporremo un ordine del giorno, che speriamo venga approvato, nel quale si invita a prevedere nella legge di stabilità per il 2014 iniziative dirette a dare stabilità all'agevolazione fiscale per l'efficientamento energetico degli edifici, così da permettere - ripeto - il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020. Negli ultimi anni, anche grazie al determinante impulso dell'Unione europea, è emersa la necessità di promuovere l'efficienza energetica dei Paesi membri considerando, oltre alle azioni specifiche sull'efficientamento energetico, la dimensione economica e sociale dello sviluppo, intesa come occasione per migliorare la competitività e la ricerca e, conseguentemente, accrescere l'occupazione e la produttività. la produttività. La definizione di indirizzi e azioni per ridurre i consumi di energia attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica e per abbattere l'emissione dei gas serra è una priorità a cui il sistema Paese deve dare risposte e indirizzi precisi e certi. Ridurre i consumi energetici è una priorità anche nell'ambito degli obiettivi 20-20-20 in materia di efficienza energetica. In particolare, nel settore edile, essi rappresentano il 40 per cento del totale di energia consumata nell'Unione europea. confronto deve essere focalizzato sullo strumento della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica degli edifici - ecobonus - che dal 2007 ad oggi ha generato numerosi benefici. Le detrazioni sono uno dei principali strumenti contenuti nella strategia energetica nazionale proprio per il raggiungimento di questi obiettivi previsti al 2020. Nel tempo questo meccanismo si è sempre più diffuso nel territorio nazionale. Nei primi cinque anni di attività, circa il 5,5 per cento del patrimonio edilizio nazionale ha subito un ciclo di riqualificazione energetica, globale o parziale, e si stima che circa il 5 per cento delle famiglie italiane abbia beneficiato della detrazione del 55

I risultati registrati nel periodo 2007-2011 sono molto considerevoli. Ci sono circa 1.300.000 pratiche totali e ci sono investimenti complessivi per 15.500 milioni di euro. Insomma, c'è un risparmio energetico complessivo di energia primaria superiore a 8 milioni di gigawattora l'anno. Diciamo che gli investimenti in edilizia di qualità, in risparmio energetico, in fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca e, più in generale, in interventi di *green* *economy* sono un importante volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, perché consentono di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività

Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, il decreto ecobonus ritorna in Senato dopo alcune modifiche sostanziali apportate alla Camera. Alcune variazioni sono però negative, come l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e approvato dalla maggioranza, che stabilisce che il certificato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. È a nostro avviso un altro errore, che segue quello legato all'emendamento, sempre del Movimento 5 Stelle, presentato qui al Senato e approvato da tutti (tranne che dalla Lega Nord), che introduce l'obbligo di rilascio dell'attestato anche agli edifici trasferiti a titolo gratuito. Dunque un'altra norma, cari colleghi, che introduce nuove incombenze e oneri a carico dei proprietari degli immobili, specie in questo particolare momento di crisi. Ma il decreto ecobonus non doveva rispondere alle attese dei contribuenti? *(Applausi si insiste nel voler fare i primi della classe alle spalle della povera gente, pur di sventolare la bandiera dell'ambientalista? Fortunatamente, però, ci sono anche importanti modifiche migliorative, come la stabilizzazione degli incentivi a partire dal prossimo anno, grazie ad un emendamento presentato dalla Lega Nord e votato - lo sottolineo - all'unanimità con il parere favorevole del Governo che vincola l'Esecutivo a superare la fase delle proroghe. Positiva l'estensione dei benefici, dopo le pompe di calore e gli elettrodomestici introdotti in prima lettura, anche alle schermature solari e alla microcogenerazione, nonché agli interventi di efficientamento idrico e di sostituzione dell'amianto, ma soprattutto all'adozione di misure antisismiche sugli edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità sismica. Sarà inoltre salutato con favore dalle famiglie l'annullamento dell'irragionevole ed incoerente previsione di aumento dell'IVA (dal 4 al 21 per cento) sui supporti integrativi ai testi scolastici *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, previsione sulla quale il nostro Gruppo qui al Senato in prima lettura aveva presentato, dopo un primo emendamento bocciato, un ordine del giorno poi sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari. Prima di concludere, voglio evidenziare, da una parte, i dubbi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine alla mancanza di risorse statali a copertura degli emendamenti migliorativi dall'altra, il ruolo del Governo, che ha invece manifestato la propria intenzione di sostenere per proprio conto gli oneri necessari alla copertura del provvedimento. Appare evidente che un simile atteggiamento denota mancanza di responsabilità da parte dell'Esecutivo, perché l'incognita sulla copertura finanziaria rischia di tradire ancora una volta le aspettative dei cittadini e delle imprese; ed è proprio quello di cui non abbiamo bisogno.

dal Gruppo LN-Aut).* Mi sembra che sia un esempio molto interessante di come si usino bene i soldi dei cittadini; quindi una pizzicatina ve la meritate, visto che siete così bravi. Detto questo, su questo provvedimento ‑ entrando nel merito ‑ è stato approvato in prima lettura un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle in cui si chiedeva di valutare un piano per efficientare tutto il patrimonio immobiliare pubblico, con un orizzonte a venticinque anni. Siccome è stato approvato questo ordine del giorno, stimoliamo il Governo ad intervenire in tal senso.

Riteniamo buono il riferimento all'esigenza di contenere il consumo del territorio; peccato che, di fatto, non vi siano strumenti che sanzionino la violazione o l'elusione della norma. In questo modo, l'articolo si limita ad esprimere una buona intenzione e nulla più. Allo stesso modo, ritengo sia stata una buona scelta quella di consentire l'utilizzo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-*ter* anche agli ospedali

conciliare l'esigenza di certificazione con la necessità di non gravare il bene primario della casa, magari scadenzando con cura i tempi di adozione della certificazione. Basterebbe usare un po' di buonsenso. due parole alla banca dati nazionale in cui far confluire i flussi dati relativi ai beneficiari. Questa è una modifica interessante, che riteniamo buona:

se vogliamo realmente intervenire su questo settore assolutamente primario, che è in crisi come tutto il settore edile, gli interventi di efficientamento possono dare una grande spinta in questo settore e, quindi, magari l'utilizzo di incentivi ci può aiutare in tal senso. Magari sarebbe anche interessante, solo sul fronte delle fonti termiche, valutare - questo magari lo chiederemo al Governo - il fatto il fatto di rendere compatibile la detrazione fiscale con i certificati bianchi. Anche questo è, infatti, un settore in crisi e le fonti termiche hanno sostanzialmente un costo molto ridotto, ma possono dare un grande contributo

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto energia torna al Senato e porta con sé il forte auspicio che gli incentivi possano stabilizzarsi per il 2014.

presentazione che dà forza a un lavoro che abbiamo fatto in Commissione, sia alla Camera che al Senato. Gli incentivi di carattere strutturale hanno riguardato l'efficienza idrica ed energetica, il sismico, la messa in sicurezza degli edifici, la depurazione delle acque inquinate da arsenico e la sostituzione delle coperture in amianto.

Rimane il problema delle piccole e medie imprese. Ultimamente anche le imprese a gestione familiare, che sono riuscite più di altre a tenere i saldi aziendali discreti, stanno cominciando ad avere dei grossi problemi.

compromettendo l'intero settore economico, rischiando di banalizzare quanto di buono c'è in questo provvedimento. Queste misure sono una sacca di sangue data ad una economia anemica.

Questo decreto-legge va comunque nella giusta direzione per quanto riguarda alcune misure in esso contenute, ma noi vigiliamo che lavoro e rilancio delle piccole medie imprese non restino solamente un'illusione. Siamo stati anche un po' critici sul sistema di

se gli va di lusso (e quando dico "gli va di lusso" vuol dire se riescono ad accedere al credito), dai 2 ai 3 punti di interesse in più rispetto a quelle tedesche quando ottengono un prestito. Questa è un'altra questione che va affrontata sicuramente In questo provvedimento ci sono cose buone e cose sicuramente migliorabili. Abbiamo aziende e imprenditori buoni, abbiamo lavoratori in gamba: in gamba: dobbiamo solo fare cose buone per loro e metterli nelle condizioni migliori per lavorare. Questo è l'auspicio del mio Gruppo su un provvedimento che sicuramente

*(M5S)*. Signora Presidente, svolgerò un intervento più breve rispetto a quello previsto, per cui le chiedo la cortesia, eventualmente, di recuperare nella fase di illustrazione degli emendamenti il tempo risparmiato. Signora Presidente, onorevoli colleghi, parlare di risparmio energetico in questo periodo va di moda. Lo ha testimoniato poc'anzi l'intervento del collega senatore Arrigoni,

nella fase cruciale che l'Italia e l'Europa attraversano - il loro apporto alle decisioni da prendere per il rinnovamento del Paese. C'è da lavorare concretamente, con pazienza e spirito costruttivo, spendendo e acquisendo competenze innanzitutto nelle Commissioni di Camera e Senato». Signora Presidente, questo non è un discorso che ho fatto io: lo ha fatto il presidente Napolitano. Noi abbiamo

Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per esprimere la massima soddisfazione del Governo nei confronti del Senato, così come abbiamo fatto alla Camera, dove abbiamo prodotto un lavoro molto

apre una nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 16-*bis*.100, mentre è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Prego

Mi scusi, signora Sottosegretario, ma non riusciamo a lavorare. Prego i senatori Segretari di ritirare le tessere dalle postazioni non occupate dai senatori.

di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico, anche il superamento dei valori limite

su cui, proprio grazie a questo strumento, abbiamo cominciato a ottenere dei risultati importanti. Lo stesso aumento della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in un momento di crisi enorme di tutto il settore edilizio, è un'opportunità per fare quell'operazione di riconversione anche delle delle piccole e medie imprese nella grande opera che abbiamo davanti a noi, ossia la riqualificazione energetica degli edifici e la rigenerazione urbana, la ristrutturazione edilizia.

rese stabili e strutturali.

in tutte le politiche energetiche, e soprattutto nelle politiche ambientali, è assolutamente fondamentale la stabilità delle misure e delle regole;

Questo per noi è assolutamente fondamentale.

anche in via generale, e introdurla anche all'interno della norma che riguarda gli incentivi per gli elettrodomestici (bastava non aggiungere la parola "grandi"). Però, anche questo è un passo che noi valutiamo positivamente.

la detrazione del 65 per cento anche agli interventi di ristrutturazione per l'adeguamento antisismico, ma tale misura è stata ristretta soltanto alle zone 1 e 2, lasciando fuori,

Monti. Abbiamo notato che si continua ad oscillare, con atteggiamenti che non sono certamente favorevoli a una strategia e ad una sovranità energetica nazionale. Ritengo sia arrivato il momento di non limitarci soltanto

complessivamente, delineando con chiarezza la strategia del Paese. Questo decreto sta a testimoniare che investire sull'efficienza energetica, sull'ambiente, sulla riqualificazione e la ristrutturazione edilizia è non soltanto un esempio di economia compatibile con l'ambiente, ma anche l'esempio di come l'ambiente possa costituire una risposta e un'opportunità importante per uscire dalla crisi in questo Paese. Per tale motivo il Gruppo Misto-SEL voterà a favore del provvedimento.

quando parla di quote latte e degli allevatori del Nord si informi prima di parlare, di dire falsità e luoghi comuni. Legga, studi la relazione dei carabinieri depositata presso tutte tutte le procure d'Italia, nella quale si dimostra che al Sud ci sono centinaia di allevatori con quote, ma senza vacche e senza latte.

all'ordine del giorno. Oggi questa Assemblea si appresta a licenziare un provvedimento che certamente in questa fase di recessione per il Paese può rappresentare un efficace strumento di sostegno ai consumi e allo sviluppo delle imprese, specie quelle del settore edile. Per questo motivo il nostro voto, lo dichiariamo fin da ora, sarà favorevole. Un voto favorevole che, tuttavia, non nasconde il nostro rammarico nel constatare come, anche in questa occasione, il Governo non abbia inteso compiere nessun passo avanti per l'adozione di una politica industriale di più ampio respiro, finalizzata a restituire competitività al tessuto produttivo del Paese. Gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno, e quindi contrastare, se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano, che è caratterizzato da piccole e medie imprese, a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia del Paese. Queste imprese sono oggi in uno stato di profonda sofferenza. Molte di loro sono ormai condannate alla chiusura a causa della scarsa liquidità di cui dispongono, dovuta alle difficoltà di accesso al credito bancario, e della forte oppressione fiscale, che è fra le più alte d'Europa. L'impresa che fallisce, non a causa di debiti ma per mancati pagamenti, specie da parte della pubblica amministrazione, non per mancanza di capacità o di spirito di iniziativa, ma per chiusura delle banche a concedere finanziamenti, incarna il fallimento dello Stato. I principali responsabili di questa crisi economica internazionale, che ha investito anche il nostro Paese, sono certamente gli istituti finanziari e le banche. che oggi, negando il credito alle imprese e alle famiglie, le condannano al fallimento e alla disperazione. Questa crisi internazionale non è un fenomeno virtuale. Esplode, infatti, in una data precisa, il 2007, con il fallimento di una delle più grandi banche d'affari americane, la Lehman Brothers. Le strategie speculative adottate da queste banche, attraverso la realizzazione di una finanza creativa, hanno causato la morte dell'economia reale. Per troppi anni abbiamo abbandonato un concetto molto elementare: dal lavoro e dall'ingegno si genera la produzione e, quindi, la ricchezza. Signori miei, il mito del re Mida di trasformare il piombo in oro era follia allora e lo è ancora di più oggi. Le stesse banche responsabili della crisi che stanno vivendo famiglie e imprese in realtà non hanno pagato e non pagheranno mai nessuna conseguenza per i loro comportamenti deviati. Gli errori del passato poco hanno insegnato: invece di sanzionare i comportanti speculativi adottati dalle banche d'affari, le stesse sono state rifinanziate e ricapitalizzate, e per giunta senza obbligarle ad evitare nuovi atteggiamenti speculativi e ad aperture al credito alle imprese e alle famiglie. Poco fa, questa Assemblea ha approvato la conversione in legge di un decreto-legge con il quale il Governo ha di fatto commissariato un'azienda privata perché ritenuta responsabile di avere causato negli anni danni all'ambiente e alla salute dei cittadini.

Quindi non dirò più "signori del Governo", che spero comunque leggeranno questo intervento, e mi rivolgerò solo alla Presidenza e agli onorevoli senatori. In questi anni gli istituti finanziari e le banche d'affari sono stati artefici di atteggiamenti che potrebbero essere ricondotti alla fattispecie di reato di istigazione al suicidio. Quanti imprenditori, privati del credito e costretti a non pagare i loro operai, si sono sentiti in colpa per aver disonorato un impegno che, con fatica, veniva portato avanti da generazioni? Non sopportando quest'onta, disperati, non hanno avuto altre soluzioni, se non togliersi la vita! La nostra non è una provocazione! Se voi, e mi riferisco ai signori del Governo, purtroppo assenti, ma qualcuno riferirà loro...

limiti alla finanza speculativa. Abbiate il coraggio di farlo guardando negli occhi i familiari delle vittime di questa crisi. E se avrete questo coraggio, signori, cosa che siamo certi non avverrà mai, vi promettiamo fin da ora la nostra fiducia e il nostro sostegno, perché dimostrereste di non essere servi della grande finanza e dei poteri ma di essere veramente al servizio del popolo! Presidente, questo decreto-legge è un'importante opportunità di crescita e di ripresa per settori in pesante difficoltà. Esso prevede la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, riallineandolo pienamente con l'Unione europea e mettendo la parola fine a due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, avviate dalla Commissione europea. Si indica un percorso chiaro e definito, finalizzato a favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, stimolare la diversificazione energetica, le fonti rinnovabili e la ristrutturazione antisismica, promuovendo, ristrutturando e migliorando la qualità del patrimonio edilizio Scelta Civica è soddisfatta dei risultati raggiunti con questo provvedimento, che contribuisce al risparmio energetico e migliora nel contempo la situazione edilizia del nostro Paese. Il decreto contribuisce quindi allo sviluppo economico e al potenziamento di una filiera edilizia e impiantistica, fatta di imprese industriali e artigianali, in cui l'Italia è attrezzata e all'avanguardia. Fra tutti gli interventi contenuti nel decreto, fondamentale è l'innalzamento della detrazione per interventi di efficientamento energetico dal 55 al 65 Altrettanto opportuno è stato prolungare a tutto il 2014 gli incentivi in questione, restando l'auspicio di Scelta Civica affinché gli incentivi stessi diventino strutturali, congiuntamente ad altri interventi che coniughino efficienza energetica, stimolo all'economia e lotta all'evasione fiscale. Se, poi, particolari benefici ne trarrà l'edilizia, che negli ultimi anni ha perso circa mezzo milione di posti di lavoro, vantaggio ne trarranno anche il legno arredo, le cucine e l'industria del bianco, settori che hanno davvero sofferto in questi anni. Ma questo provvedimento è importante perché non incide semplicemente sulla ripresa economica, ma va anche, come hanno evidenziato altri colleghi, nella direzione di tutelare le famiglie e i cittadini italiani, migliorando l'ecologia, per così dire, dell'ambiente domestico. di un decreto che si muove nella giusta direzione, tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga. Ad esempio, come già da noi sottolineato in un ordine del giorno approvato nel precedente passaggio in Senato, vanno incentivati gli strumenti di accumulazione energetica domestica e industriale, connessi all'uso di energie rinnovabili. Più in generale, le incentivazioni fiscali sono un formidabile - e, tutto sommato, relativamente poco costoso

e soprattutto la società civile italiana, intesa in questo caso come il mondo degli imprenditori, industriali e artigianali, i sindacati, il mondo finanziario ed i consumatori. Tutte queste categorie, infatti, ci chiedevano (e attendono tuttora) una stabilizzazione della normativa legislativa in merito ad un sistema di detraibilità fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e consolidamento antisismico. Dovrebbe essere una considerazione banale e scontata che imprese e cittadini hanno bisogno di un quadro normativo stabile e di lungo periodo per poter programmare, da un lato, le proprie produzioni e i propri servizi e, dall'altro, i propri acquisti di tali prodotti e servizi. Ma questa considerazione banale sembra essere un'eccezione nel nostro Paese, in generale e in questa situazione specifica in particolare, dal momento che sinora si è provveduto più e più volte a prorogare una misura incentivante di brevissimo periodo, creando quindi nella società civile italiana un atteggiamento di diffidenza, incertezza e sfiducia nelle istituzioni: sentimenti che, di fatto, si traducono in un disincentivo ad investire a lungo termine creando sviluppo economico. Preso quindi molto tristemente atto che la maggioranza del Senato non aveva saputo recepire correttamente tali istanze, che pure avevamo udito in prima persona in sede di audizione presso la 10a Commissione (la Commissione competente), proviamo ora una certa soddisfazione nel recepire quanto elaborato dai nostri colleghi della Camera dei deputati. La Camera infatti, anche grazie a una determinante azione del Movimento 5 Stelle, ha provveduto a fare un passo avanti. È un passo avanti potenzialmente e decisamente importante, in quanto si enuncia di voler rendere strutturale un regime di incentivazione fiscale e di volerlo fare entro la fine di quest'anno. quest'anno. Noi del Movimento 5 Stelle, che in questo ultimo mese abbiamo incontrato giornalmente le parti sociali interessate, vigileremo attentamente affinché questo si traduca in realtà. Lasciate però che io mi dolga fortemente del fatto che, nel corso degli incontri che abbiamo svolto come Movimento 5 Stelle con le suddette parti sociali (industriali, artigiani, sindacati, banche, consumatori), abbiamo ricevuto numerose e costanti lamentele e proteste da parte di queste, che hanno affermato di essere troppo poco ascoltate dalla politica: ripeto, troppo poco ascoltate. Infatti le parti sociali ci hanno ribadito che solo durante la campagna elettorale i soggetti politici cercano una comunicazione e l'appoggio delle parti sociali, salvo poi diminuire drasticamente la quantità e la qualità dei rapporti con le stesse nel corso della legislatura. Ebbene, noi del Movimento 5 Stelle stiamo e vogliamo continuare a procedere in maniera diversa, e continueremo a rapportarci quotidianamente con le imprese, i consumatori, il mondo bancario e i sindacati, per definire assieme la migliore politica per una ripresa economica e sociale. Vigileremo pertanto affinché le promesse vengano correttamente mantenute e proveremo a colmare le lacune dal momento che il presente decreto ne ha almeno due piuttosto importanti: la prima è che non vi è una disposizione chiara che concretizza un supporto bancario predefinito per coloro che volessero utilizzare questo strumento di detrazione fiscale. Mi sembra persino superfluo ricordare che nessuna idea è buona se non vi sono le risorse finanziarie per procedere. In questo momento molti cittadini sono in gravi difficoltà con le spese correnti; figuriamoci come possono affrontare spese straordinarie di una certa entità senza un adeguato supporto finanziario. È quindi necessario che la politica si accordi con il sistema bancario per approntare una convenzione che permetta in maniera il più possibile semplice ed automatica di accedere ad un prestito a tassi agevolati per privati che vogliano realizzare un intervento di efficientamento energetico o antisismico. Questo infatti conviene a tutti: alle banche, perché sicuramente avranno la loro parte di guadagno, come è giusto; al privato, perché potrà rifarsi con i risparmi che l'intervento di efficientamento gli procurerà nel tempo; tempo; all'intero sistema economico, perché si sviluppa produzione, commercio e servizi relativi. In questo ambito di ragionamento auspichiamo anche che il mondo bancario sappia cogliere le enormi opportunità che gli derivano dalla presenza di tutte quelle agenzie ed imprese che si occupano di progettare e realizzare progetti di efficientamento energetico senza esborso diretto da parte del cliente, dal momento che vengono ripagate da risparmio realizzato in bolletta. Anche in questo caso il Movimento 5 Stelle si è già mosso facendo partire un fattivo e costante dialogo con il mondo bancario, e continuerà a farlo controllandolo e coinvolgendolo nel dialogo con le tutte le altri parti sociali coinvolte. La seconda lacuna è l'eccessiva diluizione nel tempo del periodo di recupero dell'investimento effettuato, cioè in pratica il fatto che sono necessari dieci anni per recuperare, con il meccanismo del credito d'imposta sulla propria dichiarazione dei redditi, l'importo dell'agevolazione concessa. Anche in questo caso il recentissimo confronto con le parti sociali ci ha confermato quella che dovrebbe essere una considerazione scontata e ovvia, e cioè che molti cittadini e aziende preferiscono accordarsi su uno sconto immediato e sul fatto (ripeto, in nero: non nascondiamoci dietro una foglia di fico, per favore), con i conseguenti danni per il sistema economico e fiscale collettivo, piuttosto che dover aspettare un periodo di tempo così lungo - troppo lungo - per recuperare l'investimento. Pure in questo caso, quindi, il Movimento 5 Stelle si impegnerà per modificare la situazione; ci auguriamo che gli altri soggetti politici ci aiutino nel momento in cui si discuterà sul modo in cui rendere strutturale tale incentivo e dare facoltà a chi ha effettuato l'investimento di recuperarlo fiscalmente con i tempi a lui più consoni. Questo decreto è dunque un piccolo passo avanti e può diventare un discreto passo avanti se le promesse di stabilizzazione verranno mantenute; esso non è sufficiente per svincolarci dalla schiavitù energetica cui siamo, nostro malgrado, sottoposti. Infatti, siamo tuttora alla mercé delle fonti fossili - petrolio, gas, carbone e pertanto auspichiamo che vi sia da subito un cambiamento di politica rispetto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A chi ancora si ostina a sostenere l'argomento del costo eccessivo delle fonti rinnovabili, fornisco un solo dato per tagliare la testa al toro: la Germania - sulla cui serietà mi sembra non si possa discutere - ha calcolato in 40 miliardi di euro

quindi non direttamente all'interno della bolletta elettrica; ciò, però, chiarisce inequivocabilmente come le fonti fossili siano antieconomiche. il nostro non è un atteggiamento di estremismo ambientale, ma al contrario è un mero conto economico. L'oligopolio energetico significa, inoltre, avere pochi produttori e relativamente poca manodopera impiegata; viceversa la produzione distribuita e diffusa in migliaia di piccoli impianti comporta uno sviluppo tecnologico ed uno sviluppo del relativo indotto con ordini di grandezza del personale potenzialmente impiegato decine di volte superiori. Anche in questo caso, pertanto, parliamo di creazione di lavoro e non facciamo discorsi da talebani ambientali. In Italia abbiamo un enorme e drammatico problema di mancanza di lavoro. L'efficienza energetica e le fonti rinnovabili rappresentano una grande opportunità per creare molte migliaia di nuovi posti di lavoro: Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno calcolato in 1,6 milioni i posti di lavoro che possiamo creare fino al 2020. Il Movimento 5 Stelle, quindi, continuerà ad impegnarsi e a coinvolgere tutte le associazioni di imprenditori che - come ho già evidenziato - sono unanimi nell'approvare questa *vision* per il nostro futuro.

Penso che maggiore attenzione da parte del Ministero dell'economia avrebbe fatto guadagnare tempo.

francamente ci si mette a disagio. Tanto più che con questo ping‑pong si sono determinati - come ha fatto giustamente rilevare la senatrice De Petris - anche degli errori, perché francamente obbligare un mercato della locazione che è già in difficoltà ad allegare anche l'attestato di prestazione energetica pare una cosa abbastanza irrazionale. È stato approvato un ordine del giorno; noi francamente ci auguriamo, come Popolo della Libertà, che il provvedimento che oggi viene approvato all'unanimità venga pubblicato immediatamente sulla *Gazzetta Ufficiale* e che questo consenta a noi di porre rimedio nel decreto del fare a quello che è stato oggettivamente un errore. Fatte queste considerazioni, che faccio non per spirito polemico, ma proprio in funzione di un miglior rapporto e di una maggiore efficienza per il futuro, desidero sottolineare con grande soddisfazione il senso di responsabilità dei partiti che non appartengono alla maggioranza, proprio prendendo atto che è stato fatto comunque un cammino parziale, ma positivo, e che viene approvato oggi un provvedimento penso in via definitiva ‑ che fa del bene al Paese sia sul piano ambientale che sul piano economico. *(PD)*. Signora Presidente, signora Sottosegretario, vorrei anzitutto ringraziare i due relatori, i Presidenti delle Commissioni e tutti i membri della Commissione finanze e della Commissione industria per la celerità e la responsabilità con cui hanno affrontato in terza lettura questo provvedimento. Lo abbiamo definito già l'altra volta, in prima lettura, un primo passo importante; i temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione edilizia, accompagnati da misure fiscali a sostegno, che sono state ulteriormente consolidate nel passaggio alla Camera, non solo ci convincono,

giustamente dovrà trovare un processo di stabilizzazione attraverso nuovi interventi, a nostro parere all'interno di un quadro strategico che, come giustamente sottolineato anche dal Governo, andrà definito nei prossimi mesi, non solo in ragione delle risorse necessarie da destinarvi.

come ha detto anche lo stesso Sottosegretario durante la sua replica - erano aspetti sottolineati e sollecitati nella discussione del Senato, non solo delle Commissioni

che sono stati richiamati da noi attraverso un ordine del giorno, oppure gli interventi sulle misure antisismiche, che auspichiamo trovino future correzioni e allargamenti per includere le aree colpite di recente da eventi sismici, rappresentino un punto sicuramente importante. Da ultimo, ritengo significativo anche il fatto che alla Camera si sia provveduto a soddisfare una richiesta che nel Senato aveva trovato elementi di forte sollecitazione, ovvero il tema dei supporti integrativi: per effetto delle modifiche apportate, infatti, restano salvi dall'aumento dell'IVA gli allegati ai supporti scolastici e ai libri Per queste ragioni, ovviamente, il Gruppo del Partito Democratico voterà nuovamente a favore ed auspica - appunto - che questo primo passo sia significativo, non solo come stimolo all'economia del nostro Paese, ma anche propedeutico ad interventi più strutturali nel campo dell'efficientamento energetico

*(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, intervengo solo per un veloce ma necessario ringraziamento in terza lettura, anzitutto ai due relatori, senatori Sciascia e Tomaselli, che devo dire con gran attenzione hanno seguito un provvedimento di particolare delicatezza ed interesse. anche la sottosegretaria Vicari che, sia in prima che in terza lettura, ci è stata vicina e ha permesso quell'interlocuzione positiva. Rivolgo un ringraziamento anche agli Uffici per il lavoro ed il supporto che ci hanno dato - permettetemi, chiudo qui - alle Commissioni, perché il vero passaggio delicato è quello che si è svolto ieri nelle Commissioni riunite. Faccio riferimento a quanto detto sia dal senatore Carraro che dal senatore Rossi. Questo vuole rappresentare un auspicio per coloro che si occupano di riforme istituzionali per un ragionamento sul bicameralismo perfetto. Penso che la possibilità di una seconda lettura alla Camera dei deputati abbia permesso di introdurre delle pressanti novità che erano state richieste all'interno di quest'Aula in relazione all'articolo 19 e che hanno permesso di portare importanti e significative migliorie.

Presidente, onorevoli colleghi, vorrei segnalare la situazione che verrebbe a prodursi per effetto del decreto legislativo 7 ordine alla chiusura del tribunale di Sanremo e all'accorpamento dello stesso al tribunale di Imperia. In particolare, verrebbe meno un presidio importante del territorio che ha visto svolgersi significative inchieste relative ad attività di organizzazioni criminali. Inoltre, l'accorpamento andrebbe a creare disagi per gli utenti e per gli operatori di giustizia nel doversi recare ad Imperia, che non potrebbe svolgere, come Sanremo, funzioni di tribunale di frontiera. Infine, l'accorpamento e la chiusura del tribunale di Sanremo non produrrebbe l'auspicato risparmio di risorse organizzative, in quanto il tribunale accorpante dovrebbe comunque strutturare spazi ed uffici per adeguare il servizio, senza voler poi considerare i rischi che l'accorpamento produrrebbe in termini di cumulo di lavoro, soprattutto delle cause ancora pendenti. Pertanto, pur condividendo la necessità di procedere ad una riorganizzazione più razionale ed efficiente del sistema giustizia, chiedo al Governo di valutare più attentamente ogni singola situazione che verrebbe che verrebbe a prodursi con la nuova geografia giudiziaria.

Questa mattina, in sede di dichiarazione di voto, la senatrice D'Onghia ha affermato che qualcuno in quest'Aula racconta delle favole e parla di 1.600 morti per la città di Taranto. Poi ha paragonato questa situazione

Bangladesh, India o situazioni geografiche di questo tipo non siano tanto differenti tra loro.